Grazie L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Senatrice Russo - come da lei ricordato - la recente sentenza del TAR Lazio n. 2915 del 2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3409 del 2018, si è pronunciata per l'annullamento della nota del 15 maggio 2017, contenente indicazioni agli uffici scolastici regionali sull'organico del personale docente, in particolare sulla ripartizione delle ore di insegnamento di strumento musicale. Al riguardo si precisa che la nota oggetto di ricorso per l'anno scolastico 2017/2018, per la parte impugnata, ha esplicitato quanto già definito nel pertinente decreto interministeriale relativo all'organico docente, e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione, in coerenza con il contenuto della relazione tecnica al regolamento n. 89 del 2010, in cui viene ribadito che l'insegnamento (esecuzione e interpretazione) è impartito dedicando il tempo del docente a due o tre alunni, per una media di 2,5 alunni per ora docente. Inoltre, le sentenze sopra richiamate sono intervenute per tale disciplina (classe di concorso A-55 *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016), ritenendo che l'esigenza di contenimento della spesa, come disposto dall'articolo 64

Pertanto, secondo tale giurisprudenza, per le lezioni di primo strumento musicale va garantita agli alunni un'ulteriore ora frontale per l'apprendimento tecnico-pratico al primo biennio. Occorre anche considerare che l'attuale schema di decreto interministeriale per l'anno scolastico 2018-2019 ricalca il precedente dell'anno scolastico 2017-2018, in quanto è stato elaborato e trasmesso per il previsto concerto del MEF prima delle più recenti pronunce giurisdizionali, con la conseguenza di aver già dispiegato i propri effetti sulle connesse e complesse procedure di mobilità e di immissione in ruolo. Alla luce di quanto sopra esposto, la soluzione prospettata dalla senatrice interrogante di ricalcolo del nuovo organico e modifica delle graduatorie di mobilità non è praticabile per l'anno scolastico 2018-2019, in quanto gli effetti di un tale intervento sarebbero incompatibili con il regolare proseguimento dello stesso anno scolastico. In conclusione, vorrei chiarire che da parte di questo Ministero vi è la concreta intenzione di superare le criticità evidenziate dalla senatrice interrogante con la massima celerità e soprattutto con una soluzione che sia davvero efficace, ciò tenuto anche conto del parere dell'Avvocatura generale dello Stato pervenuto nei primi giorni di luglio, in cui si suggerisce di tenere in debita considerazione il principio di diritto enunciato nelle pronunce giudiziali in occasione dell'adozione dei prossimi provvedimenti. Questo potrà avvenire solo attraverso ponderati ed adeguati interventi anche di natura normativa, che potranno consentire l'aggiornamento dei quadri orari ordinamentali dei licei musicali. Tale azione sarà effettivamente in linea con la giurisprudenza di merito e al tempo stesso comporterà un effettivo ampliamento dell'organico per l'anno scolastico 2019-2020, compatibilmente in ogni caso con le risorse finanziarie disponibili.

annuncio che mi ritengo soddisfatta della risposta fornita. Sottolineo che la questione affrontata è stata affrontata dal precedente Governo, che, con una semplice nota ministeriale, aveva illegittimamente disapplicato la legge, come già dichiarato più volte dalle sentenze. Non posso quindi che accogliere con soddisfazione la notizia che si è deciso di invertire la rotta, di tutelare il diritto allo studio e di ottemperare alle sentenze. Mi auguro però che quanto riferito possa essere attuato il prima possibile per garantire così non solo il diritto allo studio dei nostri ragazzi, ma anche la qualità dello studio stesso in un contesto internazionale molto competitivo,

Signor Presidente, colleghi senatori, per quanto riferisce la società ANAS, il progetto definitivo della strada statale 372 Telesina relativo all'adeguamento a quattro corsie dal chilometro zero al chilometro 60-900 è suddiviso in un primo lotto dal chilometro 37, svincolo di San Salvatore Telesino, al chilometro 60-900, svincolo di Benevento (approvato dal proprio consiglio di amministrazione in data 20 novembre 2017), e da un secondo lotto, dal chilometro 0-A1 Caianello al chilometro 37, svincolo di San Salvatore Telesino, per il quale è in fase di avvio una specifica gara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Per il primo lotto, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione, la società ha avviato la procedura per la localizzazione e per la dichiarazione di pubblica utilità, con la trasmissione dei relativi atti progettuali a tutti gli enti interessati. Il 15 dicembre 2017 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha convocato i Comuni e la stessa ANAS per la presentazione del progetto. Successivamente al parere del predetto Consiglio, il progetto definitivo, corredato dei pareri degli enti interessati, è stato presentato al CIPE dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione, per la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità. Nella seduta del 28 febbraio 2018, il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'intervento. Nelle more della registrazione presso la Corte dei conti e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE, sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo per l'appalto dei lavori, che si prevede possa concludersi entro il mese di dicembre 2018 con la pubblicazione del bando di gara. In risposta al secondo, al terzo e al quarto quesito posto, ANAS informa che, al fine di eliminare i dissesti causati dalle eccezionali condizioni meteorologiche del mese di febbraio scorso, sono stati eseguiti ripristini provvisori lungo la strada statale in argomento. Inoltre, ANAS ha programmato un ulteriore intervento, finanziato e già appaltato in regime di accordo quadro, finalizzato al risanamento della pavimentazione stradale, in tratti saltuari, per un investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro; successivamente saranno riesaminati i limiti di velocità nei tratti interessati dall'intervento. Per quanto riguarda la segnaletica stradale, quella esistente risulta rispondente alle esigenze del tracciato e alle vigenti prescrizioni del codice della strada, in applicazione dei princìpi di chiarezza e di essenzialità che la segnaletica deve assicurare. Quanto all'eventualità di interdire il transito dei mezzi pesanti, ricordo che la strada statale 372 è una strada extraurbana e, pertanto, idonea al transito anche dei suddetti veicoli. In ogni caso, ricordo che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono disciplinati annualmente i divieti di circolazione fuori dai centri abitati per particolari categorie di veicoli di trasporti stradali, in alcuni giorni e orari, in occasione di giornate in cui è previsto maggior traffico.

che ho sottoscritto insieme ai colleghi Lonardo e De Siano, sulle gravi condizioni in cui versa la strada statale 372 Telesina. Ci tengo a precisare che i settanta chilometri in questione rappresentano il principale collegamento da e verso Roma per la provincia di Benevento e il territorio di Caserta e altresì collegano Benevento a Caianello e, quindi, all'autostrada A1. Si tratta, La Telesina ha un tratto di strada a solo due corsie che versa in condizioni non adatte alla tipologia di traffico intenso, anche di mezzi pesanti, che quotidianamente veicolano sulla strada statale. Il manto stradale risulta ancora ad oggi disconnesso, nonostante l'ANAS avesse indetto, nel non troppo lontano 2016, un bando di gara per il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale. Centinaia di migliaia di cittadini attendono da anni che il progetto di raddoppio delle corsie venga finalizzato, ma ancora una volta pare si dovranno rassegnare a promesse e a tempi sicuramente ancora lunghi. L'ultimo impegno politico su questa infrastruttura risale al 2009, quando il Governo Berlusconi, attraverso lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro dal CIPE, realizzò una serie di importanti infrastrutture in Regione Campania con il varo del piano nazionale delle infrastrutture strategiche per il triennio 2009-2011; un impegno finanziario che consentì allora la realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo regionale, a partire dal raddoppio della superstrada Benevento-Caianello, fino al collegamento tra la tangenziale di Napoli alla rete stradale e al servizio che porta alla costiera amalfitana. Avevamo chiesto al Governo di conoscere quali misure intendesse adottare per migliorare e intensificare la segnaletica stradale in alcuni tratti inesistente o non adeguata;

pulita sono gli investimenti che l'Italia aspetta e merita. Oggi prendiamo atto del fatto che le nostre domande rimarranno inascoltate e che nessuna misura adeguata sarà adottata. Ancora una volta prendiamo atto del fatto che questo Governo non tutela l'incolumità degli automobilisti. Parlando a nome di quei cittadini che ogni giorno percorrono decine di chilometri, posso tranquillamente affermare quanto in questo momento siano sconsolati dalla superficialità che l'Esecutivo sta dimostrando. Sembra che sulle infrastrutture questo Governo stia brancolando nel buio: non ha la forza di mettere in campo un piano di azione serio in tema di infrastrutture, manutenzione e soprattutto sulla messa in sicurezza del nostro Paese. Ovviamente, per spirito di Patria, stendo un velo pietoso su come il Governo sta gestendo l'emergenza a Genova, con un estenuante balletto di decreti, nomine commissariali, *boutade* ministeriali che hanno prodotto fino ad ora soltanto un risultato: quasi due mesi di chiacchiere.

Signor Presidente,per fornire una compiuta risposta al quesito posto dall'interrogante è doveroso ricordare la *ratio* sottesa al decreto legislativo n. 149 del 2015, per mezzo del quale si è deciso di istituire un'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. Occorre in questa sede ricordare che l'istituzione dell'Agenzia non ha comportato il passaggio nei suoi ruoli dei funzionari ispettivi di INPS e INAIL, i quali invece sono formalmente rimasti, per espressa previsione dello stesso decreto istitutivo dell'Ispettorato medesimo, alle dipendenze dei rispettivi istituti. Ciononostante, l'inquadramento professionale dell'ispettore del lavoro è destinato in prospettiva a diventare unico, atteso che le nuove assunzioni di ispettori del lavoro potranno essere effettuate, in base al dispositivo normativo, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Ciò premesso, non corrisponde al vero il fatto che il personale INPS ed INAIL non è impegnato nell'attività ispettiva, con ciò che ne deriverebbe - ad avviso dell'interrogante - in termini di omesso contrasto a fenomeni intollerabili come quello del caporalato che, al contrario, rappresenta un tema centrale per il Ministero che oggi rappresento. È doveroso invece evidenziare che, proprio in considerazione della diversità degli assetti organizzativi e gestionali del personale ispettivo di diversa provenienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha posto in essere una serie di attività volte a uniformare e valorizzare le competenze di tutto il personale ispettivo. È stata quindi svolta un'intensa attività di formazione rivolta al personale dell'INPS e dell'INAIL avente a oggetto le funzioni di polizia giudiziaria, l'esercizio del potere di sospensione dell'attività imprenditoriale e l'utilizzo della diffida accertativa quale strumento per tutelare i crediti da lavoro dei dipendenti. Viceversa, per il personale ispettivo già dipendente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati avviati e definiti specifici percorsi formativi in materia previdenziale e assicurativa che, oltretutto, non hanno comportato ulteriori oneri per l'amministrazione, essendo stati organizzati avvalendosi delle strutture e del personale dell'Ispettorato e degli istituti. Attraverso tale attività è stata dunque garantita una maggiore uniformità di competenze che, in prospettiva, consentirà una maggiore fungibilità del personale di vigilanza e, quindi, di poter impiegare con maggiore efficacia tutto il personale ispettivo verso obiettivi che, di volta in volta, costituiscono una priorità d'intervento, così come già avviene in relazione al fenomeno del caporalato. L'avviso manifestato dall'interrogante è che una reale programmazione dell'attività ispettiva sul territorio possa fare a meno delle commissioni territoriali di programmazione, definite addirittura inutili. La convinzione che sorregge l'azione del Governo è di implementare tutte quelle misure intese a responsabilizzare il maggior numero di soggetti istituzionalmente coinvolti nella vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. In tale prospettiva va in questa sede ricordato che, ferma restando l'individuazione delle linee di intervento da parte della commissione centrale di coordinamento della vigilanza, presieduta dal Ministro del lavoro, l'istituzione delle commissioni regionali di coordinamento ha consentito, su quasi tutto il territorio nazionale, di procedere a una selezione degli obiettivi di vigilanza più significativi, in relazione ai fenomeni territorialmente più rilevanti, consentendo di evitare la sovrapposizione degli interventi ispettivi, seppur sporadici. È proprio nell'ambito di tale programmazione a livello territoriale che sono stati condivisi appositi progetti di vigilanza speciale, quale quello per il contrasto al caporalato, posto all'attenzione dall'odierno interrogante. Per quanto concerne l'attività di vigilanza in materia di caporalato principalmente, ma non esclusivamente nel settore agricolo, desidero evidenziare che la stessa è stata implementata e sollecitata in più occasioni e che sono attualmente in corso numerosi accessi ispettivi che prevedono la movimentazione di personale ispettivo da tutta Italia verso quegli ambiti territoriali dove si concentra maggiormente il fenomeno. Un'efficace azione repressiva richiede infatti, in primo luogo, le disponibilità di un congruo numero di unità di personale ispettivo che, laddove possibile, deve essere affiancato da personale militare. In tal senso voglio rappresentare che l'Ispettorato si avvale del fondamentale supporto sia della Guardia di finanza che dell'Arma dei carabinieri. Proprio questi ultimi, infatti, oltre ad operare nell'ambito di ciascun Ispettorato territoriale del lavoro, cosiddetto Nuclei ispettorato lavoro (NIL), e nell'ambito di ciascun Ispettorato interregionale del lavoro, cosiddetti Gruppi

per i rispettivi ambiti di competenza, tutti i livelli di Governo, centrale e territoriale, nonché il personale civile e militare, quale unica via che consentirà di poter debellare queste odiose situazioni di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera connesse a fenomeni di caporalato.

buon auspicio il lavoro che state conducendo verso la figura dell'ispettore unico e verso l'obiettivo di fungibilità delle figure presenti che abbiano un'uguale competenza a livello nazionale. Ciò non toglie che, a livello di sussidiarietà, vediamo un'eccessiva vicinanza al territorio, vediamo ledere il principio di efficienza ed efficacia dell'azione e quindi, ancora una volta, vi invitiamo a tener presente la nostra segnalazione, evitando inutili, dispendiosi ed eccessivi nuclei di vicinanza al territorio che potrebbero essere sostituiti dagli ispettorati esistenti.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Noi, invece, da lei oggi ci aspettiamo una sola frase: «Restituiamo i soldi che abbiamo portato via ai comuni cittadini;

con immediati e successivi atti del Governo e, dunque, decreti. Lo stesso *Premier*, tra l'altro, aveva anche citato in quale provvedimento avrebbe inserito il rifinanziamento: rifinanziamento: il decreto per la sicurezza. Ora di tutto ciò non c'è traccia. Ministro, noi ci aspettiamo che il Governo abbia parole di verità. Dicevo poc'anzi che, quando non si sa cosa dire, si dice di tutto e il Governo ha detto di tutto per nascondere questo taglio vergognoso dei soldi alle periferie, ai cittadini più disagiati e al recupero delle nostre città. era stato sbloccato l'avanzo di amministrazione e che, dunque, questi soldi avrebbero sostituito il finanziamento per le periferie, ma sappiamo benissimo che questo non c'entra nulla. Lo sa meglio di me. L'avanzo di amministrazione - come ribadito da una duplice sentenza della Corte costituzionale - rappresenta risorse dei Comuni; invece, il bando delle periferie è finanziato con soldi dello Stato. Si è parlato di incostituzionalità, ma lei sa benissimo che la sentenza della Corte costituzionale stabilisce una parziale incostituzionalità per un terzo del finanziamento e la stessa sentenza dice che è sanabile - ciò rientra nella sua competenza diretta - attraverso la convocazione della Conferenza unificata con i presidenti delle Regioni. Bastava inserire il tema per il 6 settembre o discuterne il 20 settembre nella Conferenza da lei presieduta e la parziale incostituzionalità sarebbe stata radicalmente superata.

e dunque nel fatto che un po' alla volta ci si dimentica di questi soldi promessi. Ancor meno vogliamo immaginare che ci sia nel Governo qualcuno che immagini

ascolteranno la sua risposta centinaia di sindaci e soprattutto i venti milioni di cittadini che hanno diritto a questi finanziamenti.

Il decreto-legge milleproroghe ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni con 96 Comuni, Capoluogo di Provincia o Città metropolitana, con riguardo al programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto sono destinati a un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione L'effetto primario della disposizione è quindi una redistribuzione delle risorse tra tutti gli enti che hanno prodotto avanzi di amministrazione. Tra di essi vi sono anche alcuni dei 96 enti per i quali è stata differita l'efficacia delle convenzioni in essere. Devo puntualizzare che tale modifica legislativa è stata introdotta in quest'Aula tramite un emendamento d'iniziativa parlamentare con il voto favorevole di tutti i Gruppi. La situazione di incertezza normativa si è determinata - come sapete - a seguito della nota sentenza n. 74

Non è possibile qui ricordare i caratteri problematici che la sentenza ha individuato rispetto ai connotati del fondo di cui all'articolo 140. Basti qui rammentare che la Corte ha fatto salvi i procedimenti di spesa in corso, laddove si possa determinare altrimenti un pregiudizio di diritti costituzionali

la sede e il momento dell'intesa; la ricognizione dei procedimenti afferenti a materie di competenza regionale; la ricognizione dei procedimenti in corso; il monitoraggio degli interventi e della congruità effettiva delle risorse.

Rimane ferma per gli enti la possibilità di procedere in autonomia con riguardo agli interventi per i quali sono previste anche risorse derivanti dal cofinanziamento, ovvero di accendere forme di anticipazione finanziaria nei limiti consentiti. In ogni caso il Governo, in ragione anche degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio, intende adottare specifiche misure destinate alla legge di bilancio 2018 per garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti. Nel frattempo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha adottato, proprio ieri, un'apposita circolare per consentire l'immediato utilizzo per spese di investimento degli avanzi. Per quanto riguarda la Conferenza unificata, faccio presente che, in qualità di Presidente, avevo inserito, su richiesta delle Regioni, ANCI e UPI, nell'ordine del giorno del 27 settembre, l'intesa sul ma la Conferenza non ha potuto dare un'intesa su un provvedimento già pubblicato in Gazzetta e che scaturisce da una norma che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima nella parte in cui non prevede le intese. Ricordo che la sentenza della Corte non ha nemmeno specificato se era necessaria l'intesa e pone quindi in dubbio tale

Ho provato a invitare il Presidente dell'ANCI a ripensare a tale forma di protesta, che invero produce effetti anche di blocco nei confronti di altri provvedimenti d'interesse di Regioni, Province e degli stessi Comuni.

gli avanzi significa infatti sbloccare dei soldi dei Comuni ma qui stiamo parlando di soldi che aveva messo lo Stato per fare investimenti importanti nelle periferie. Credo che ciò sia veramente paradossale e che siamo di fronte ad una situazione che continua a non essere definita. State facendo il gioco delle tre carte sulla pelle dei Comuni, dei cittadini e dei luoghi che devono essere riqualificati. Questo è inaccettabile e il PD non farà cadere nel dimenticatoio questa situazione: saremo sempre qui

con il decreto dignità sono stati reintrodotti, in una veste diversa rispetto alla disciplina precedente, i cosiddetti *voucher*. Tuttavia con la nuova disciplina è stata introdotta anche una serie di nuovi adempimenti, che ne rendono complicato l'utilizzo, in particolare per le imprese agricole. L'INPS non ha ancora fornito indicazioni chiare sulla loro applicazione e sul suo sito la procedura è farraginosa e difficilmente utilizzabile. Prima dell'utilizzo è necessario il versamento del compenso sul conto virtuale, ma la cifra viene accreditata in media solo dopo dieci giorni e prima non è utilizzabile. Inoltre, dalla nuova disciplina sono escluse quelle aziende agricole che superano il limite di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non a caso i rapporti attivati, a differenza delle esperienze precedenti, sono solo poche decine di migliaia, decretandone così il sostanziale fallimento. Vi è poi il caso degli enti locali, che per assicurare i servizi socio-assistenziali in condizioni eccezionali e temporanee si avvalgono di cooperative sociali e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e che oggi lamentano l'assenza di uno strumento burocraticamente semplice per garantire l'erogazione dei servizi menzionati. Per tutte queste ragioni, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno reintrodurre l'istituto dei *voucher* così come era prima della loro abrogazione, avvenuta con il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, reintroducendo gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e di voler inserire tra i possibili beneficiari anche persone iscritte regolarmente nell'assicurazione generale obbligatoria. Si chiede altresì di sapere se non sia possibile estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che organizzano, anche per conto dei Comuni, i servizi sociali, assistenziali e socio-pedagogici.

un uso improprio dello strumento, a scapito di forme di lavoro più stabili. Il decreto dignità limita l'ambito di applicazione dei *voucher* alle imprese del settore agricolo, alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori e ha ampliato anche per gli enti locali l'arco temporale di utilizzo delle prestazioni occasionali, da tre a dieci giorni. I *voucher* possono essere utilizzati per far lavorare titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni (se regolarmente iscritti a un ciclo di studio, anche universitario), disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno del reddito. Devono anche risultare non iscritti, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il decreto dignità ha inoltre previsto alcune semplificazioni tra cui la nuova modalità di pagamento del lavoratore che si aggiunge a quelle esistenti. Quanto alla possibile estensione dell'utilizzo delle prestazioni occasionali agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, vorrei precisare che l'attuale disciplina non impedisce di far ricorso alle prestazioni occasionali, purché lo si faccia nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e del divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. *(Applausi Signor Ministro, la sua è stata una mera spiegazione del testo che conosciamo benissimo. Abbiamo sentito poco di nuovo, devo dire, nella sua risposta. Comunque

Non sono state individuate le coperture necessarie alla proroga della mobilità e allo sblocco dell'*iter* relativo al pagamento delle precedenti annualità. anche attraverso una dialettica con la Regione Lazio, il problema si è concentrato sulla mancanza di 5 milioni e mezzo di euro. tutto questo non è sufficiente a risolvere le criticità di quest'area, però è anche chiaro che è assolutamente necessario che vengano portate a conclusione le procedure per la sottoscrizione dell'accordo di programma e la pubblicazione dei bandi per la reindustrializzazione dell'area. La seconda questione, Ministro, sulla quale credo che si siano già tenuti alcuni incontri al Ministero dello sviluppo economico, riguarda la vertenza relativa alla Unicoop Tirreno che vede centinaia di lavoratori rischiare il proprio posto a causa di un piano industriale sbagliato che prevede la cessione, tra l'altro, degli otto punti vendita del Sud del Lazio.

Signor Presidente, prima di tutto voglio ribadire la disponibilità, che ho dato anche ai rappresentanti dei lavoratori e ai segretari dei vari sindacati, sulla questione che che riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga che dovranno essere rinnovati perché abbiamo centinaia di migliaia di persone che rischiano di restare senza reddito perché ad un certo punto, nel 2015, si è scelto di accorciare la durata della cassa integrazione. Quindi, in generale, tengo prima di tutto a dire che non solo siamo molto sensibili a questo tema ma sono contento del fatto che alle quattro della scorsa notte grazie alla reintroduzione della cassa integrazione per cessazione del cosiddetto decreto emergenze, abbiamo evitato che oltre 300 persone finissero in mezzo alla strada nella vertenza Bekaert. Adesso troveremo il *partner* per reindustrializzare quello stabilimento. Per quanto riguarda invece lo stato di crisi che ha investito il gruppo Coop Italia e l'attuale situazione del piano industriale di razionalizzazione e dismissioni, abbiamo seguito le iniziative dei sindacati, preoccupati per le gravi ripercussioni socioeconomiche che potrebbero derivare dall'attuazione del piano industriale dell'Unicoop Tirreno, contenente la cessione di otto punti vendita, come diceva lei, nel Sud del Lazio. Al tavolo, in presenza di tutti, l'azienda ha descritto una situazione generalizzata di crisi e di perdite costanti soprattutto negli otto punti vendita citati, che si vorrebbero dismettere. Il Ministro dello sviluppo economico, con la condivisione dei partecipanti al tavolo, ha chiesto ai rappresentanti dell'azienda di bloccare il percorso avviato di cessione dei punti vendita, di avere dall'azienda in tempi brevi una risposta circa l'inizio di un percorso di confronto unitario e condiviso con le parti sociali e l'intervento, alla prossima riunione del tavolo ministeriale, del presidente e del direttore generale di Unicoop Tirreno. Una cosa è certa: questa crisi non vogliamo sottovalutarla, ci sono tante famiglie coinvolte. Con la pratica ormai rodata dell'ascolto attento dei lavoratori, sono sicuro che arriveremo a una soluzione che possa soddisfare gli interessi di tutti, come tanti altri tavoli che abbiamo chiuso negli ultimi mesi*.

all'azienda di sospendere la cessione e la chiusura dei punti vendita. Ovviamente contiamo sul fatto che sul punto si continuerà a essere determinanti, anche perché vorrei ricordare a lei - e anche a me stessa - che

di pubblica, consolidata e diffusa conoscenza la problematica degli elevati prezzi dei carburanti e dei servizi di ristorazione lungo la rete autostradale nazionale,

divario talmente significativo da non potersi in alcun modo ritenere motivato da fondanti ragioni di mercato. È noto che i concessionari delle tratte autostradali impongono agli operatori cui viene affidato il servizio di vendita *royalty* elevatissime - per quanto riguarda i carburanti, sui volumi erogati e, per quanto riguarda la categoria *food and beverage*, sui valori delle vendite - che gravano sulla formazione dei prezzi di vendita ai consumatori,

5 miliardi di euro e ciò si accompagna anche ad un aumento molto elevato dei nostri pedaggi autostradali che, come lei ben sa, Ministro, sono i più alti d'Europa. conto di tutto questo e considerando che l'imposizione delle *royalty* da parte dei concessionari nei termini che ho descritto sopra costituisce di fatto una modificazione peggiorativa delle condizioni, sia per quanto riguarda i consumatori, ma anche per quanto riguarda quelle aziende che operano con i rischi sulla propria pelle e sui propri investimenti, le chiedo, Ministro, quali urgenti iniziative intende adottare alla luce delle criticità evidenziate in premessa, al fine di verificare la correttezza la correttezza della condotta di imporre *royalty* e assicurare in ogni caso condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato senza effetti distorsivi per le imprese

Grazie Presidente e grazie a lei, senatrice. Il tema della correttezza dell'imposizione di *royalty* nelle concessioni dei servizi autostradali, tra i quali quelli connessi ai carburanti o alla ristorazione, non può prescindere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: si discute, infatti, della gestione delle concessioni autostradali. Il ruolo del Ministero dello sviluppo economico in questo ambito è definito con decreto interministeriale MIT-MISE del 2015, in cui è stato approvato un piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali che viene aggiornato ogni cinque anni e che prevede una revisione straordinaria su richiesta motivata del concessionario e del concedente solo in caso di eventi straordinari. Per quanto riguarda le *royalty*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva espresso la preferenza per la loro determinazione in valore fisso, specificando che lo si poteva fare per massimizzare i volumi di vendita e per ridurre l'impatto del canone, con contestuale diminuzione del prezzo e/o miglioramento della qualità. L'Autorità aveva anche ipotizzato un possibile sistema misto alternativo e l'adozione nei bandi di gara di meccanismi di revisione dei prezzi, in modo da consentire l'adeguamento della *royalty* fissa a parametri oggettivi (per esempio, la variazione di flussi di traffico sulla rete autostradale). Stiamo lavorando insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per trovare tutte le possibili soluzioni al problema. In generale, però, voglio ricordare che il nostro Governo si è impegnato a rivedere tutto il sistema si è impegnato a rivedere tutto il sistema delle concessioni, da quelle autostradali a quelle delle acque minerali. È diventato chiaro agli occhi di tutti, con il drammatico crollo del ponte di Genova, che il sistema attuale non funziona; non si può quindi andare avanti in questa maniera. Lo Stato deve essere più presente ed esercitare maggiori funzioni di controllo sul concessionario, in particolare quando ne va della sicurezza e della vita dei cittadini. Là dove poi ci siano stati degli abusi, è ovvio che la stessa concessione possa essere ridiscussa. Nel decreto emergenze abbiamo stabilito che la società Autostrade non ricostruirà il ponte, grazie ai poteri straordinari di cui è dotato il commissario, la cui nomina è stata ufficializzata oggi. A questo voglio fare gli auguri di buon lavoro al nuovo commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, il sindaco Marco Bucci. Adesso Governo centrale e amministrazioni locali hanno gli stessi oneri, le stesse responsabilità e una grande sfida da vincere insieme: risollevare Genova. *(Applausi Signor Ministro, non posso essere soddisfatta della sua risposta. Intanto mi sembra una risposta

gli auguri al sindaco Bucci, il nuovo commissario, perché credo che finalmente, dopo tanto tempo, Genova e tutta l'Italia possano avere uno spiraglio di luce e il famoso ponte. Però mi dispiace dirle, signor Ministro, che nel decreto-legge emergenza nulla di quanto le ho chiesto ho visto rappresentato; invece, mi sembra che sui cittadini abbia un impatto davvero molto forte. avrei dovuto chiedere al ministro Toninelli, ma lei mi risulta anche essere Vice *Premier* di questo Governo. Comunque, a parte le parole poco soddisfacenti, mi auguro che lei ci sappia sorprendere tutti con i fatti e le auguro buon lavoro. *(Applausi dai

festeggiato l'abolizione della povertà - così avete detto - grazie al reddito di cittadinanza. L'avete festeggiato dal balcone, come da molto tempo non succedeva, e credo che nessuno lo rimpiangesse

Poi ieri sera, lei stesso, ministro Di Maio, ha chiarito su Facebook che un miliardo, di quei 10 miliardi, serve per potenziare i centri per l'impiego e solo 9 miliardi vanno ai cittadini assistiti. Ne prendiamo atto. Questa mattina, l'altro Vice Presidente del Consiglio, il ministro Salvini, ha dichiarato che in realtà per il reddito di cittadinanza e tutto il resto ci sono solo 8 miliardi in tutto, dunque compreso il potenziamento dei centri per l'impiego. Ma, ministro Di Maio, io mi schiero con lei, nel senso che prendo per buona la cifra che lei stesso, poche ore fa, alle 20,30 di ieri, ha detto: 9 miliardi. E farò anche conto che si tratti di soldi nuovi, e cioè non magari provenienti dal reddito di inclusione o da altre forme di assistenza, altrimenti

Fatti i conti, sa quanto viene a testa al mese per questi 9.368.000? Esattamente 80 euro, anzi 80 euro e 6 centesimi. Insomma, il Governo del cambiamento, le feste sul balcone e sul barcone, le liti a livello internazionale che si sono già costate 3 miliardi di maggiori interessi che ci siamo già impegnati a spendere in più sul debito pubblico, per avere i soliti 80 euro? È una misura che voi avete criticato, e anche noi, perché la ritenevamo inadeguata, illusoria e costosa. Lei ha detto, però, che sarà solo per 6,5 milioni di cittadini. Ma allora vuol dire che 2.868.000 italiani poveri non vedranno un centesimo da questo reddito di cittadinanza? Feste solo per voi e non per loro? Quanto ai 6,5 milioni di presunti fortunati, si tratta di 115 euro al mese, perché dobbiamo dividere i soliti 9 miliardi - Salvini permettendo - per 6,5 milioni: fa 115 euro al mese. Ma come, abbiamo tutti imparato a memoria la magica cifra dei 780 euro al mese, e poi al momento buono sono solo 115? Signor Ministro, il problema della legge di bilancio è che la si fa con i numeri e non con gli annunci, e i conti devono tornare, come ben sanno tutte le famiglie italiane. ringrazio il senatore Malan, che voglio prima di tutto rassicurare: ci sono i fondi per realizzare tutte le misure della legge di bilancio; ce ne sono così tanti che ripaghiamo pure i debiti di quelli che c'erano prima, infatti l'IVA non aumenta. per questa interrogazione, perché mi dà la possibilità di spiegare come funziona il reddito di cittadinanza, che è prima di tutto una misura di politica attiva del lavoro. al lavoro per rilanciare prima di tutto i centri per l'impiego: lo stiamo facendo con collaborazioni con università degli Stati Uniti e con un confronto con il Governo tedesco, infatti lunedì vi sarà un incontro tra me e il Ministro del lavoro a Berlino. Ovviamente, il reddito di cittadinanza si rivolge, come diceva lei, senatore Malan, a persone in stato di povertà relativa e in stato di povertà assoluta. C'è prima di tutto un dettaglio che bisogna tener presente: le persone in stato di povertà relativa non sono a zero ed è questo che non torna nel conto - lo dico senza polemica - che faceva lei. Il reddito di cittadinanza vuol dire che a tutti deve essere garantito un reddito di 780 euro vincolato a: lavori di pubblica utilità; formazione continua durante la giornata; non rifiutare più di tre proposte di lavoro. questo non vuol dire che a tutti andranno 780 euro. Se una persona, per esempio, ha un reddito di 500 euro, ne percepirà 280 se entra nel programma di riqualificazione e formazione e lavori di pubblica utilità; se una persona ha un reddito di 200 ne percepirà 580; chi ha reddito zero percepirà 780 euro. Poi, la platea di cui parla lei è fatta anche di stranieri e non di cittadini italiani lungosoggiornanti e noi abbiamo ristretto il reddito alla platea dei cittadini italiani lungosoggiornanti Quindi, mettendo insieme la decurtazione del numero dei 10 milioni e il fatto che non tutti prenderanno 780 euro ma sarà un reddito integrativo a quello che già si guadagna,

è una misura che non dà un solo euro a chi se ne sta sul divano, perché tutti dovranno avere la giornata impegnata per la formazione e per i lavori di pubblica utilità. Questo vuol dire anche che i beneficiari non avranno il tempo di lavorare in nero e, se imbrogliano, si beccano fino a sei anni di galera per dichiarazioni non M5S e L-SP-PSd'Az).* Quindi, abbiamo inserito in questa norma anche una serie di misure che contrastano i furbi, perché noi ci vogliamo rivolgere solo alle persone perbene, a quelle che si comportano onestamente. *(Applausi mi permetta di dire che questa manovra, che noi abbiamo chiamato "manovra del popolo", è una manovra rivoluzionaria perché, finalmente, ripaga il popolo dopo che per anni il popolo italiano ha dovuto pagare sprechi, privilegi, pensioni d'oro, vitalizi, Air Force Renzi, e chi più ne ha più ne metta. per ora gli italiani hanno ripagato voi con milioni di voti, che indubbiamente avete preso, ma facendo conto sulle vostre promesse, che mi sembra si stiano sempre più allontanando rispetto a quanto state facendo. 115 euro a testa per solo circa due terzi dei poveri credo non sia davvero quello che gli italiani si aspettavano. Certamente, ha ragione lei: non tutti i poveri sono a zero, ma tanti lo sono. Sa a quanti bastano 780 euro? Bastano per 961.000 persone: ci sono 780 euro al mese per 961.000 persone, con quei 9 miliardi per i quali lei ci ha assicurato che ci sono le coperture. Allora, io credo che gli italiani si aspettassero qualcosa di parecchio diverso, il problema, come lei ha detto, è che i conti bisogna farli tornare. La media è quella, per cui ci saranno forse delle limitazioni. Concludo citando Umberto Bossi, che proprio stamattina ha detto che l'assistenzialismo non ha mai risolto i problemi di questo Paese, e citando Milton Friedman, che ha detto: se pagate chi non lavora e tassate chi lavora (lei addirittura ha detto che se uno lavora - giustamente, per carità - e prende il reddito di cittadinanza va in galera per sei anni), difficilmente creerete altro che disoccupazione.

premesso che il recupero occupazionale è il punto cardine della riforma dei centri per l'impiego e del reddito di cittadinanza, misura di proattività volta a restituire dignità ai lavoratori ed ai cittadini in generale, appare necessario favorire il più rapido reinserimento dei lavoratori nel circuito occupazionale ponendo in essere, a tal fine, azioni formative e di supporto al reddito mirate, che rispondano ad un'attenta analisi e corrispondenza precisa tra domanda e offerta di lavoro di lavoro dei diversi territori. Considerato che, a causa di erronee politiche attuate dai precedenti Governi, un gran numero di lavoratori sta perdendo il proprio posto di lavoro, rischiando conseguentemente di restare senza reddito, attualmente presso il Ministero dello sviluppo economico risultano attivati circa 160 tavoli di crisi aziendale che coinvolgono circa 180.000 lavoratori, particolare attenzione deve essere riservata alla situazione delle imprese che cessano l'attività, ma appaiono in grado di garantire la continuità occupazionale e produttiva in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda a soggetti terzi. Si chiede pertanto di sapere quali azioni il Governo intenda porre in essere per venire in aiuto dei lavoratori delle imprese citate, al fine di non disperderne il patrimonio aziendale comprensivo delle risorse umane, garantendo altresì la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori interessati. delle politiche sociali*. Signor Presidente, a mio parere le politiche sul lavoro portate avanti precedentemente in questi anni hanno devastato i diritti dei lavoratori e non hanno portato alcun significativo vantaggio alla nostra piccola e media impresa; anzi, gli imprenditori sono stati contemporaneamente soffocati dalla burocrazia e dal fisco. Non parlo per sentito dire, ma perché tutti i giorni, nel ruolo che rivesto, sono tenuto ad ascoltare i problemi delle vittime di questa politica scellerata.

quando ce n'è bisogno, con la mia persona. Lì ci sono i problemi reali delle persone, da lì derivano le risposte ai bisogni veri dei lavoratori e degli imprenditori. Anche grazie a questo confronto abbiamo deciso di reintrodurre, come ho detto, con il decreto-legge emergenze, la cassa integrazione per cessazione, che ci sta consentendo di dare un futuro e una prospettiva di lavoro a migliaia di famiglie che non vivranno di cassa integrazione. Si tratta, infatti, solo di una misura ponte in attesa della reindustrializzazione di siti che cessano di funzionare perché qualcuno, qualche prenditore, qualche multinazionale decide di andarsene in Romania o in Polonia e di lasciare oltre 300 famiglie in mezzo ad una strada. La scelta di eliminare questa tutela con il *jobs act* è stata assolutamente folle e sarebbe bastato sedersi a parlare con i lavoratori per non farlo; evidentemente, si preferiva parlare solo ed esclusivamente con lobbisti e banchieri. *(Applausi dai Gruppi M5S e ed è per questo che portiamo avanti la grande riforma dei centri per l'impiego, che è il punto cardine su cui poggia l'introduzione del reddito di cittadinanza. Se da un lato bisogna inserire nel mondo del lavoro i giovani, spesso disorientati e sconfortati dalle difficoltà nel trovare la prima occupazione, dall'altro il nostro Governo è vicino e sta lavorando per le migliaia di lavoratori che dal 24 settembre scorso hanno iniziato a non avere più la cassa integrazione straordinaria. Infatti, stiamo elaborando una serie di norme e di provvedimenti per ripristinare questi strumenti in tempi brevi. Non lasceremo nessuno da solo, lavoratori e imprenditori. Non lasceremo che nessuno finisca

Signor Ministro, io posso ritenermi soddisfatta della sua risposta. Accogliamo con favore l'introduzione di questo strumento che mira, ancora una volta, a dimostrare come questo Governo e questa maggioranza stiano proseguendo proseguendo il cammino a fianco dei cittadini e soprattutto dei lavoratori, ma non solo, anche degli imprenditori, che negli ultimi anni sono stati mortificati da politiche poco attente ai loro bisogni effettivi. Questo non lo diciamo noi, riceviamo ogni giorno *feedback* dai cittadini

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo intervento desidero riportare la nostra memoria ad un tragico evento di cui ieri ricorreva il settimo anniversario. Alle ore 12,21 del 3 ottobre 2011 un drammatico crollo di una palazzina scosse il centro urbano di Barletta, coinvolgendo emotivamente l'intera Italia. Maria Cinquepalmi, Antonella Zaza, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Tina Ceci, quattro giovani lavoratrici di un opificio posto al piano terra della palazzina, e la figlia quattordicenne del titolare del laboratorio, rimasero sepolte sotto le macerie del crollo e persero la vita. A loro il nostro ricordo, ai loro cari il nostro rinnovato cordoglio. Altre due donne, di cui una al quinto mese di gravidanza, furono invece estratte vive dalle macerie, con un'ardita, commovente e memorabile impresa dei Vigili del fuoco, dei quali essere sempre fieri. Come acclarato nei giudizi penali, fino alla recente sentenza del grado d'appello, il tragico disastro fu causato da varie imperizie nei lavori che si stavano eseguendo accanto al palazzo crollato, per demolizione e ricostruzione di un edificio. Eppure, erano stati avvertiti e denunciati vistosi segni premonitori. È incredibile che, nell'epoca in cui si misurano spostamenti millimetrici tra i continenti, non siano state eseguite le collaudate indagini del caso. Le cause indirette del crollo, non giudicabili in processi penali, ma censurabili da un punto di vista sociale, culturale e politico, sono da imputare ad una frequente pessima gestione dell'edilizia urbana. Squarciare un agglomerato urbano vecchio di oltre un secolo è un'operazione sempre pericolosa. Meglio la salvaguardia, a beneficio della sicurezza e della conservazione del patrimonio edilizio storico e architettonico di pregio. Si devono privilegiare piani di recupero dei centri storici rispetto a sostituzioni edilizie o a nuovi piani di espansione urbana. Il degrado del centro storico è anche frutto delle spropositate colate di cemento periferiche, che coagulano deleteri interessi intrecciati e consumano scelleratamente suolo. Fermare il consumo di suolo, rilanciando il patrimonio edilizio esistente e favorendo programmi di rigenerazione urbana è un imperativo del contratto per il Governo del cambiamento. Onore alle vittime e siano esse un monito estremo per scongiurare altre simili

ha visto il cedimento di una piazzola di sosta della superstrada E45 in provincia di Arezzo, all'altezza del Comune di Pieve Santo Stefano. La notizia è che il crollo ha portato alla luce la presenza di amianto in quantità quasi tre volte superiore rispetto a quanto consentito dalla legge. È questo uno dei risultati - forse il più eclatante - emerso dalla relazione tecnica consegnata in questi giorni alla procura di Arezzo. I dati provenienti dai campioni analizzati parlerebbero di ben 3.470 milligrammi per chilo di amianto presenti sul terreno prelevato dal sito. Il limite ammesso per legge però è di 1.000 milligrammi, pertanto in quel terreno ci sarebbe stata una concentrazione del 250 per cento superiore al limite consentito. Dalla cronaca si viene a conoscenza che i primi sospetti erano emersi già lo scorso marzo: a meno di un mese dalla frana, a ridosso di Pieve Santo Stefano (tra le uscite Pieve Santo Stefano Nord e Pieve Santo Stefano Sud), fu infatti sequestrata anche l'area dove il materiale era stato stoccato, mentre i lavori di risistemazione della piazzola proseguivano. Il procuratore Roberto Rossi aveva aperto un fascicolo ipotizzando il reato di disastro colposo. Secondo gli ambienti investigativi, sotto la piazzola non c'era solo terreno di riporto o roccia, ma erano presenti anche rifiuti speciali. I sospetti avanzati dalla procura di Arezzo e dai Carabinieri forestali del gruppo ambiente della procura, incaricati di svolgere le indagini, avrebbero trovato importanti riscontri. Lo studio attento e dettagliato è stato eseguito dallo studio Boeri di Livorno. Per intenderci, è lo stesso che ha svolto accertamenti nella cosiddetta terra dei fuochi e sul caso Moby Prince. Di fatto, questa presenza massiccia è la certificazione, se ancora ce ne fosse stato bisogno, del fatto che i riporti di terreno e rocce da scavo sotto quella strada sono in realtà un misto di terre e rifiuti da demolizione, e chissà cos'altro. Tutto sembra essere la certificazione che alcuni di coloro che hanno realizzato quell'arteria così importante nel corso di decenni lo abbiano fatto senza troppi scrupoli e guidati dal proprio interesse personale più che da quello pubblico. Si tratta di un indizio grave del fatto che chi avrebbe dovuto controllare l'andamento dei lavori o non lo ha fatto o lo ha fatto poco e male. Mi auguro che su questo tema si possa intervenire subito con un atto urgente o un'indagine conoscitiva per capire la situazione attuale dell'autostrada. In ambito regionale, i nostri consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini per l'Umbria ed Elisa Montemagni per la Toscana, si sono già attivati depositando una mozione al riguardo. Una volta istituita la Commissione bicamerale sugli ecoreati, chiederemo che venga aperta un'indagine e vengano anche verificati più tratti stradali, considerato che non si conosce in quanti chilometri della superstrada E45 il composto contenente rifiuti pericolosi sia stato utilizzato. La sicurezza dei cittadini, anche alla luce di recenti e tragici fatti di cronaca, deve avere la priorità assoluta: è necessario che sia fatta chiarezza, così da poter accertate ogni responsabilità. apre una nuova finestra"). Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea NATO i senatori: Cristiano Anastasi, Massimo Candura, Andrea Cangini, Alessandra Maiorino, Riccardo Nencini, Fabrizio Ortis, Adriano Paroli, Emanuele Pellegrini, Roberta Pinotti. Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della stessa delegazione i deputati: Matteo Luigi Bianchi, Edmondo Cirielli, Paolo Formentini, Luca Frusone, Luigi Iovino, Luca Lotti, Marco Minniti, Andrea Orsini, Michele Sodano.